Onorevoli colleghi, prima di passare all'ordine del giorno, la Presidenza, anche a vostro nome, saluta la delegazione della Commissione affari dell'Unione europea del Parlamento dell'Estonia, in visita di studio presso il Senato su invito della nostra Commissione per le politiche dell'Unione europea. In particolare, i colleghi parlamentari estoni sono a Roma per approfondire il tema cruciale del controllo di sussidiarietà e proporzionalità delle proposte comunitarie, alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Signora Presidente, è la terza volta in questa legislatura che alla Lega, propone in Senato mozioni dai contenuti esplicitamente antiambientali, che chiedono al Governo di mettere in discussione o di rinnegare la partecipazione dell'Italia allo sforzo della comunità internazionale, e in particolare allo sforzo dell'Europa, per fronteggiare il problema dei cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo delle energie pulite. Il pretesto di queste iniziative è sempre lo stesso: autoproclamarsi autorità scientifica e inventare una presunta incertezza della scienza su fenomeni come il *global warming*, che certo la scienza deve continuare a studiare, ma su cui esiste oggi una base di evidenze largamente condivise. Io non so perché accada tutto ciò, se per ragioni di sotterranee polemiche interne alla maggioranza (qualcuno vi ha letto il tentativo di indebolire ulteriormente il ruolo già non rilevantissimo dell'attuale Ministro dell'ambiente, testimoniato peraltro anche dalla sua assenza oggi in Aula) o per una visione del tutto paradossale delle funzioni del Parlamento, in base alla quale uno dei compiti di noi legislatori sarebbe di sovrapporci al lavoro, alle conclusioni - sempre provvisorie, ma talvolta decisive - della ricerca scientifica. So invece che, già in passato, tali prese di posizione hanno creato un forte imbarazzo al nostro, al vostro Governo, che, almeno sul piano degli impegni formali, dal G8 dell'Aquila fino alla Conferenza di Copenaghen, è rimasto ancorato agli orientamenti ed alle scelte della comunità internazionale. Ricordo che proprio a Copenaghen il ministro Prestigiacomo impiegò parecchio del suo tempo a spiegare ai suoi colleghi di tutto il mondo come fosse possibile che il Parlamento italiano votasse a maggioranza documenti dai contenuti - mi si passi l'aggettivo - così surreali. L'imbarazzo del Governo è palpabile anche in questo passaggio parlamentare. In un caso ha indotto, forse per distrazione o per errore, la sottosegretaria Ravetto ad esprimere parere negativo su uno dei punti del dispositivo della mozione che ha come primo firmatario il senatore Rutelli che si limitava a trascrivere letteralmente una parte del documento conclusivo del G8 dell'Aquila, di cui il nostro Paese, il nostro Governo, e presumo anche questa maggioranza, condividono i contenuti. caso ha costretto la stessa sottosegretaria Ravetto ad informare i firmatari della mozione presentata dal PdL e dalla Lega che non esiste alcuna clausola di revisione del pacchetto 20-20-20 chiesta ed ottenuta dall'Italia quando esso venne approvato, ormai un anno e mezzo fa. So anche - lo dico a chi oggi rappresenta il nostro Esecutivo che a me e al mio Gruppo non piace affatto l'atteggiamento scelto dal Governo per tirarsi fuori da questo evidente impaccio: far finta di niente, lasciar passare tale mozione sapendo che poi non se ne terrà nessun conto. conto. Noi preferiremmo che le parole del Parlamento, in questo caso del Senato, venissero prese sul serio e che, una volta pubblicamente condivise, fossero poi applicate. Glisso sulla visione un po' megalomane che emerge dal testo della mozione che ha come primo firmatario il senatore D'Alì, nel quale si dà sostanzialmente mandato al Governo italiano di rovesciare le decisioni dell'ONU e dell'Unione europea.

di De Boer sono di alcune settimane antecedenti il deposito della mozione del PdL. Mi fermo invece sul cuore del testo proposto da PdL e Lega, cioè sulle polemiche di questi mesi su alcuni errori, Panel on Climate Change*), che dimostrerebbero che i cambiamenti climatici sono una bufala. Peccato che, a polemiche già largamente in campo, proprio in occasione della Conferenza di Copenaghen, dove pure non si è riusciti a siglare un nuovo trattato sul clima, sia stata raggiunta per la prima volta un'intesa larghissima che riconosce la gravità del problema, la sua origine in cause legate all'uomo, la necessità di fronteggiarlo con urgenza. Ricordo a tutti i colleghi e a me stesso che vede coinvolti anche grandi Paesi come gli Stati Uniti, la Cina, l'India, che fino a pochi mesi fa avevano sempre rifiutato anche soltanto di riconoscere la gravità di questa minaccia. E peccato che, come hanno ribadito più volte le istituzioni scientifiche più autorevoli - cito per tutte l'*International Council for Science* (ICSU), che riunisce le principali accademie scientifiche del mondo, nessuno degli errori attribuiti all'IPCC

tali cambiamenti sono, in buona parte, imputabili al forte e continuo aumento delle emissioni di gas a effetto serra legate ad attività umane; se le emissioni non verranno ridimensionate in tempi brevi, la temperatura media crescerà rispetto ai livelli preindustriali di oltre 2 gradi e questo comporterà danni sociali, economici ed ambientali devastanti. Per questo, come hanno dichiarato nel loro più recente incontro i presidenti americano Obama e francese Sarkozy, la lotta al *global warming* è per la comunità internazionale una delle più decisive missioni di pace. A me dispiace che al senatore Fluttero dia fastidio l'etichetta di negazionista, ma questo è l'aggettivo usato in tutto il mondo per definire la posizione di chi, in buona fede (come sono certo nel caso suo e dei colleghi del PdL che propongono questa mozione), nega quello che viene chiamato consenso scientifico, che siano i negazionisti dei cambiamenti climatici o coloro - e ce ne sono - che rifiutano l'idea dell'evoluzione delle specie. Il Governo, dunque, di fronte alle asserzioni negazioniste contenute nella mozione che discutiamo oggi, alza le spalle e fa finta di niente, deciso probabilmente a non tenerle in alcun conto. Ma il contenuto della mozione del PdL, seppure non influirà direttamente sulle posizioni internazionali del nostro Paese, resta politicamente eloquente, poiché simboleggia bene il profilo bassissimo - uso un eufemismo - tenuto sui temi ambientali dalla destra italiana, che in questa materia cammina con una velocità velocità inferiore e talvolta in controtendenza rispetto al resto dell'Europa, e non solo. Abbiamo approvato, più di un anno fa, il pacchetto 20-20-20, ma siamo quasi gli unici a non aver ancora predisposto un piano dettagliato con la r*oad map* per raggiungere il 17 per cento di energia prodotta con fonti rinnovabili entro il 2020. Abbiamo fermato le politiche pubbliche d'incentivo al miglioramento dell'efficienza energetica, bloccando i finanziamenti per le agevolazioni fiscali a chi ristruttura la propria abitazione, migliorandone il rendimento energetico. Mentre inseguiamo l'improbabile obiettivo di un ritorno al nucleare, promettendo irrealistici e futuribili sconti sulle bollette energetiche pagate dalle famiglie, qui ed ora le famiglie italiane dovranno pagare, *pro quota*, le multe per gli sforamenti delle emissioni delle troppe centrali riconvertite a carbone. E mentre nel mondo tutti i Paesi industrializzati per uscire prima e meglio dalla crisi puntano forte sulla *green economy,* sull'innovazione energetica, sulle produzioni a basso impatto ambientale (come ha detto di recente Joseph Stiglitz, se anche non ci fosse il riscaldamento globale le azioni necessarie a contrastarlo resterebbero utilissime per il benessere futuro dell'umanità), da noi la destra continua a immaginarsi nel cuore del secolo scorso, proponendo come principale arma anticiclica la *deregulation* edilizia dell'ultimo piano casa.

sulla mozione che ha come primo firmatario il senatore D'Alia. So che la mozione presentata dal PdL verrà approvata e so che poi rimarrà lettera morta. morta. Se potessimo, voteremmo contro due volte: la prima per difendere la dignità del Parlamento, che se dà indicazioni al Governo deve essere ascoltato; la seconda per difendere il ruolo internazionale e anche il futuro sociale ed economico dell'Italia, destinati a perdersi se rimarremo nelle retrovie di un mondo in così rapida trasformazione. Signora Presidente, in prima battuta vorrei precisare la nostra posizione su alcuni passaggi importanti del dibattito di questa mattina. Innanzitutto ringrazio il Governo, in particolare la sottosegretario Ravetto, per le puntualizzazioni e le condivisioni espresse sulla mozione del PdL nella sua stragrande parte. Motiverò in seguito il perché di alcune remissioni all'Aula.

un'estensione al 30-30-30, sulla base dei risultati di Copenaghen. È in base a questo che, nel Vertice italo-francese di alcuni giorni fa, il presidente Berlusconi e il presidente Sarkozy hanno condiviso una nota inviata al presidente Barroso nella quale si impegna lo stesso Presidente a non proporre questo tipo di estensione. Lo consideriamo politicamente un primo importante passo - e dirò di questo più avanti - per una revisione, che è quella che noi proponiamo, dell'Accordo 20-20-20 nella sua interezza. Vengo al punto di maggiore critica, forse, da parte dell'opposizione riguardo alla posizione del Gruppo, supposta come in antitesi alla posizione del Governo. Non è assolutamente così. Il Governo italiano ha dimostrato in questi due anni di volere in più occasioni recuperare gli effetti assolutamente negativi di una determinazione presa da altri Governi, pur nel rispetto degli accordi internazionali che vincolano il nostro Paese. Ma se il Parlamento in questo caso - perché in altri 100.000 casi vi siete espressi in maniera diversa - non è nella possibilità di suggerire al suo Governo ulteriori azioni di modifica di accordi internazionali da altri assunti, allora siete voi stessi che negate al Parlamento di poter adottare atti di indirizzo nei confronti del Governo. In tal senso comprendo perfettamente la posizione del Governo che, là dove noi entriamo nel vivo di questa discussione invitandolo a rivedere alla radice l'Accordo 20-20-20, si rimette all'Aula perché, alla luce degli attuali accordi internazionali, è chiaro che esso non può recepire immediatamente questa proposta. Ma è altrettanto chiaro che il Parlamento la può esprimere e la può validare con il suo voto, ed è per questo che convintamente voteremo la proposta del PdL,

il verbo in materia di ambientalismo e non si rendono conto che è il loro fondamentalismo ad essere ormai fuori dai tempi; non si rendono conto che valanghe di iniziative, di *report* di stampa provenienti da tutto il mondo hanno dimostrato che il fondamentalismo ambientalista, basato sul catastrofismo - ormai è agli atti - è clamorosa impostura complessivamente proposta ai Governi da alcuni pseudoscienziati interessati a promuovere le loro personali consulenze con le grandi multinazionali piuttosto che non a indirizzare i Governi verso vere ed utili

che ancora una volta indichi la strada corretta della diplomazia internazionale perché in sede ONU si possano promuovere alcune revisioni di questi meccanismi che si sono rivelati agli occhi del mondo,

perché così entra anch'essa nel vivo e nel merito della questione. Al di là delle barriere ideologiche che si vogliono alzare ancora una volta da parte della sinistra su questi temi, chiediamo di scendere nella concretezza delle politiche ambientali,

ai grandi accordi sull'emissione di CO2, ammesso che possano risolvere il problema del cambiamento climatico, che va visto più sotto il profilo dell'adattamento che non sotto quello del più generico contrasto o della più generica velleitaria lotta. Davvero crediamo ancora che il globo possa essere gestito dall'uomo come un termosifone il cui radiatore possa essere aumentato di due o tre gradi o di mezzo grado o che debba bruciare? Mi sento un po' riportato ai tempi degli *autodafé* della Santa inquisizione quando, sotto questi profili, si voleva promuovere la purificazione dello spirito attraverso la bruciatura del corpo. *(Applausi dal Noi dobbiamo incidere sui fenomeni veri dell'inquinamento del globo (sulla deforestazione, sull'inquinamento marino, sugli inquinanti chimici) con azioni concrete che siano realizzabili. pensiamo veramente che le grandi potenze emergenti che devono sviluppare la loro economia possano adeguarsi a una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera per procedere quindi a un fermo del loro travolgente sviluppo economico? Gli inglesi, maestri di colonialismo, vogliono applicare il loro colonialismo tradizionale attraverso la politica energetica e bloccare così la globalizzazione e lo sviluppo dei Paesi emergenti. Si intervenga piuttosto sulle pratiche! Oggi ho sentito qualcuno che pure invocava il trasferimento di tecnologie. Noi siamo ben lieti di trasferire le nostre più sofisticate tecnologie ai Paesi emergenti, ma certamente non possiamo più credere che siano emergenti Paesi che ormai acquistano le nostre industrie su tutto il territorio continentale oltre che nazionale, per non dire in tutto il mondo. Allora si intervenga,

perché è stato negoziato contro gli interessi nazionali: l'Italia è il Paese più penalizzato, perché lo ha sottoscritto anche in assenza delle modalità di produzione energetica che avrebbero potuto

che le conclusioni dell'IPCC vadano sottoposte a un'analisi attenta, ad una rivalutazione puntuale, perché non è un caso che il suo Presidente sia anche consulente di 30 società multinazionali che sono orientate a sfruttare al meglio le decisioni dell'IPCC e le restrizioni che vengono imposte ai Paesi produttori di energia. Non è un caso - ripeto - che nel marzo di quest'anno

meno a rimorchio di politiche precedenti. Ho citato la politica inglese, e potrei citare quella tedesca. Vi siete chiesti come mai la Germania sia interessata all'espansione di alcuni prodotti industriali per progettare grandi campi di cattura dell'energia solare, senza però poi assumersi i rischi della gestione? Il nostro Paese deve essere più presente

questa mattina il Governo ha espresso parere contrario sul primo e sul quinto capoverso del dispositivo, rimettendosi all'Aula sulle restanti parti. Relativamente alla mozione n. 262, dei senatori Della Seta ed altri, il Governo si è rimesso all'Assemblea sul dispositivo, ad eccezione del primo, del quinto e dell'undicesimo capoverso, su cui ha espresso parere contrario. merito alla mozione n. 264, dei senatori Rutelli ed altri, il Governo si è rimesso all'Aula sul dispositivo, ad eccezione dei capoversi primo, terzo e decimo, sui quali il parere è contrario. Infine, sulla mozione n. 266, dei senatori D'Alia ed altri, l'Esecutivo ha espresso contrarietà sui primi tre capoversi del dispositivo e si è rimesso all'Aula sul restante.

ho consegnato questa mattina alla Presidenza le modifiche al testo del dispositivo della mozione n. 248, motivandole con i fatti intercorsi tra la presentazione della mozione e la discussione odierna. Oggi pomeriggio ho accolto l'invito del Governo a chiarire, premessa, cosa il Governo italiano abbia sottoscritto nel dicembre 2008 a Bruxelles, cioè una clausola, da esso stesso promossa, di dell'Accordo 20-20-20 in relazione ad alcune proposte che vi erano state, volte ad aumentare quelle percentuali al 30-30-30, cosa già fatta in prima battuta, come ho già detto, nell'incontro al Vertice italo-francese tra il presidente Berlusconi e il presidente Sarkozy, condivisa un'ipotesi di non aumento.

Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Colleghi, per cortesia!

che il presidente del Consiglio Berlusconi ha rivendicato come un successo del Governo e della diplomazia italiana. Abbiamo quindi fatto notare al Governo l'incongruità non solo del dichiararsi contrario ad alcuni paragrafi che, come ho detto stamattina, sono letteralmente uguali gli impegni che questo Governo ha assunto nell'ambito della cooperazione internazionale su queste materie,

così come c'è una posizione della Camera dei deputati, finisce per determinarsi una terza ancor più originale posizione del Senato della Repubblica. Mi chiedo: Mi chiedo: la sottosegretario Ravetto o chi altri fosse delegato dal Governo ad andare a rappresentare le posizioni dell'Italia, a quale di queste tre posizioni finirebbe per conformarsi? Si tratta di una questione che mette in una certa difficoltà, lo capisco; addirittura il Governo ha ritenuto di rimettersi all'Aula per la posizione della sua maggioranza, quindi, non ha espresso parere favorevole, mi corregga Presidente, sulla posizione della maggioranza. Conseguentemente, signora Presidente, per questi fatti molto significativi - non dal punto di vista procedurale ma

e volentieri con i firmatari la accordiamo, e concerne il penultimo paragrafo della nostra mozione, quello che inizia con le parole "a promuovere la collaborazione internazionale". Quindi, ci sarebbe una votazione per parti separate su richiesta dei colleghi dell'IdV su questo penultimo capoverso della mozione.

dando un tributo alle popolazioni colpite dal terremoto e prosegue occupandosi dei grandi temi dell'economia internazionale, della corruzione e della cooperazione internazionale e si dilunga molto, perché era all'ordine del giorno del G8, sulla questione del clima.

dispositivo di questa mozione. Sinceramente, colleghi, mi chiedo come sia possibile che oggi il Senato della Repubblica possa sconfessarle votando contro. Ultima notazione, signora Presidente, e ho finito: è evidente che, se il Senato si trasforma in un organismo parascientifico che si occupa di confutare le tesi degli uni

degli impegni e dei pronunciamenti che l'Italia ha assunto a livello internazionale. Altrimenti il risultato che ne scaturisce quale sarà? Quest'anno, Presidente, ci troveremo a dover tirar fuori come Paese oltre 850 milioni di euro derivanti dal fatto che l'Italia sconfessa gli impegni internazionali in materia di *emission trading* e, allo stesso tempo, non ha la capacità di trovare il consenso internazionale per modificarli. Il Senato, quindi, si trova ad essere l'ambasciatore di una posizione minoritaria perdente, che costa alla Repubblica italiana

Così come noi siamo preoccupati per quello che abbiamo sottoscritto e apprezziamo il lavoro semplice, umile e ossequioso sugli accordi che il Governo sta portando avanti, siamo ancora più preoccupati per quello che si potrebbe

c'è una richiesta di votazione per parti separate che riepilogo per essere chiari. Il senatore Rutelli ha chiesto che si votino per parti separate i capoversi primo e terzo del dispositivo, su cui il Governo ha dato parere contrario.

PD)*. Ho chiesto solamente una precisazione.

Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime poi parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.0.6, 3.0.8 e 3.0.9 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

e dunque introdurrebbe una norma impropria, un precetto verosimilmente non eseguibile e comunque non corretto.

sia che si tratti del primo fondo sia del secondo, introdotto con la legge del 2003 - e l'impegno del Governo a favorire il ricongiungimento familiare per coloro che sono vittime di tratta, rappresentano una precisa risposta non soltanto alla Convenzione di Varsavia, ma anche alla raccomandazione del 10 marzo 2010 del Parlamento europeo, che specificamente prevede che, nei confronti delle vittime di tratta, si debbano adoperare tutte le misure e le risorse possibili perché siano protette e assistite, anche in un percorso di recupero lavorativo, e perché nei loro confronti ci si adoperi per il ricongiungimento familiare.

ha sempre avuto una posizione d'avanguardia, sia per quanto riguarda il riconoscimento

stanziamento di risorse, che non sono illimitate, e al cui comparto di problemi già il Governo ha dedicato cospicui investimenti (come sarebbe facile ricostruire su più normative che, in filiera, si pongono nello stesso ordine logico)

altro è approvare anche il modo con cui si approvvigionano. Non so se il Governo nella sua visione strategica complessiva è d'accordo nel reperire queste risorse secondo i mezzi e le poste con cui gli onorevoli senatori indicano l'approvvigionamento. Ecco perché non è che ce ne laviamo le mani. Infine, è valutazione squisitamente politica da parte del Governo stabilire se nelle politiche politiche dell'immigrazione, per un verso, e della tutela dei soggetti che chiedono ricovero, per l'altro, queste siano finalità da considerare prioritarie nell'impiego delle limitate risorse.

mi rimetto al parere del Governo.

ribadisco qui - che in linea di massima, nel momento in cui si ratificano convenzioni, sarebbe poco opportuno che in questa sede ne approfittarne per metter mano al codice penale, perché gli interventi sul codice penale difficilmente possono essere varati in una visione organica in occasione della ratifica di una convenzione. Quindi la sede non sarebbe quella ideale. Tuttavia, al di là di questa osservazione (peraltro vi invito a non sottovalutarla), è stato già compiuto in sede di Commissione uno sforzo e un avvicinamento non lieve di posizioni, che non va tanto a merito mio o del senatore Compagna quanto del Governo stesso,

prevede di intervenire sugli articoli 600, 601 e 602 in materia di circostanze aggravanti, contemplando proprio quella casistica di aggravanti che accoglie una visione, che è nostra di maggioranza ma anche dell'opposizione, esternata in quella sede. La formula che il sottosegretario Caliendo ci ha indicato sintetizza quelle esigenze. Concludo dicendo - e non è un supplemento di replica - che la maggioranza e il Governo sono stati tutt'altro che insensibili su questo tema, se è vero che il reato stesso è stato introdotto da questa maggioranza e da un Ministro appartenente a questo Governo; quindi, la nostra parte si è in qualche modo già fatta carico dell'esigenza di adeguare l'ordinamento a questa nuova emergenza di carattere criminale. abbiamo già dimostrato con questi due fatti importanti, (l'introduzione della norma e questa formula che, pur in sede anomala, il sottosegretario Caliendo ci ha proposto, e che abbiamo tutti approvato) di aver recepito l'esigenza di modificare e rafforzare le previsioni del codice penale. Oltre non credo si possa andare utilmente e per questa ragione, che ho ritenuto di motivare, propongo agli onorevoli presentatori di ritirare i loro emendamenti. In caso diverso sarei costretto ad esprimere... Se volete che dia un supplemento di motivazione io non manco di argomenti; vedo però che non mi incoraggiate, e allora dico che, se non fossero ritirati, esprimerei parere contrario su tutti gli emendamenti.

perché prevede il rilascio di un permesso di soggiorno ai collaboratori di giustizia ammessi a programmi di protezione ai quali - tra l'altro - è già consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per fini di giustizia su richiesta dell'autorità giudiziaria. Un permesso di soggiorno *ad hoc* per i collaboratori di giustizia non può avere come effetto anche quello di consentire il ricongiungimento familiare, che si ricollega normalmente alla titolarità di permessi di soggiorno connotati da una tendenziale stabilità sul territorio, nonché al possesso di determinati requisiti di reddito e alla titolarità di un alloggio. Per la motivazione

Signora Presidente, i diritti umani sono patrimonio e conquista dell'umanità e devono trovare corpo e tutela nelle istituzioni di tutti i Paesi del mondo. La Dichiarazione universale dei diritti del 1948 ha sancito il principio della difesa della dignità degli esseri umani come obiettivo primario da conseguire nell'ambito delle relazioni internazionali e oltre gli spazi della sovranità dei singoli Stati. L'Italia ha sempre prestato molta attenzione e sensibilità nei confronti della difesa dei diritti umani e dei diritti delle persone, tanto che la Costituzione, all'articolo 2, recita come segue: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». La tratta degli esseri umani, che sia per sfruttamento sessuale o per motivi di lavoro, è una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Per questa ragione va combattuta nella duplice ottica della repressione nei confronti dei trafficanti e del supporto e della protezione sociale delle persone sfruttate. Il quadro normativo italiano in materia di tratta degli esseri umani è tra i più avanzati. Tuttavia, fino ad oggi, a distanza di cinque anni dalla firma, l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione in materia sottoscritta a Varsavia nel 2005. Oggi si colma finalmente questo ritardo. La peculiarità principale della Convenzione è che essa identifica e denuncia il disvalore proprio del delitto di tratta nella grave violazione che esso determina nei diritti fondamentali e in particolare della dignità, libertà e incolumità psicofisica della vittima. In tal senso essa non si limita a mettere in campo misure volte a contrastare il *trafficking*, ma si propone di tutelare i diritti delle vittime secondo un approccio non discriminatorio, prevedendo un efficace sistema di assistenza delle stesse. Il nostro Paese ha subito negli anni un incremento del fenomeno della tratta e le cause sono da ricercarsi nelle condizioni in cui versano i territori di provenienza delle vittime, realtà prostrate dalla povertà, ove dilaga la disoccupazione, dove le risorse sono carenti e non tutti vi possono accedere. Molte delle vittime della tratta sono state rapite da bande internazionali, altre sono state vendute dalle proprie famiglie o adescate con false promesse di lavoro. Il fenomeno è legato alla malavita organizzata su larga scala, che ricava enormi profitti dallo sfruttamento di esseri umani ed è spesso coinvolta in altre attività criminali, quali il traffico di droga e di armi. La maggior parte delle vittime proviene oggi dalla Nigeria, dai Paesi dell'Est e dall'America latina. In genere esse sono private di ogni diritto fondamentale, non dispongono di uno *status* giuridico e sono ridotte, attraverso minacce e maltrattamenti, ad una condizione di estrema dipendenza dai loro aguzzini. La tratta di persone e la schiavitù rappresentano infatti le facce di una stessa medaglia. Le donne ed i bambini sono i soggetti più esposti a questa forma contemporanea di schiavitù, basata specialmente sullo sfruttamento sessuale. Le donne sono le più soggette a diventare vittima e questo è dovuto a diversi fattori, quali la caratterizzazione al femminile della povertà, le discriminazioni di genere, nonché il *gap* di opportunità professionali esistenti nei Paesi di origine. La tratta si declina in molti aspetti. Il crimine riguarda il traffico di sesso e di lavoro, il commercio degli organi e, più in generale, qualsiasi forma di prevaricazione che sfrutta il corpo ed il lavoro delle donne, degli uomini e dei bambini. A fronte di questa situazione, solo un approccio integrato può rivelarsi proficuo per combattere la tratta di esseri umani. Il nostro Gruppo condivide I suoi obiettivi sono la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, sia in ambito nazionale che internazionale,

la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno alle stesse, sia per ragioni umanitarie sia per consentire la cooperazione con le autorità; la previsione di responsabilità penali, civili e amministrative delle persone giuridiche per un reato di tratta; la cooperazione tra autorità pubblica, organizzazioni non governative e membri della società civile al fine di prevenire la tratta e proteggere le vittime; la necessità di condurre campagne di sensibilizzazione verso le potenziali vittime. Nel dichiarare quindi il voto favorevole del mio Gruppo, voglio esprimere l'auspicio che l'occasione della ratifica della Convenzione serva anche all'Esecutivo per meditare su tali temi e sugli effetti della propria politica migratoria.

a questo strumento normativo che ratifica la Convenzione fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, che affronta in maniera decisa e concorde tra i diversi Paesi europei il gravissimo fenomeno della schiavitù

però è ancora più profondamente immorale ed offensiva per l'uomo e per la sua libertà, perché è la schiavitù del bisogno, è la schiavitù della mancanza di lavoro, è la schiavitù dell'uomo che si deve offrire, anche a rischio della propria vita, ed è trattato come merce. Quindi, pur avendo una legislazione abbastanza avanzata rispetto agli altri Paesi, sicché abbiamo dovuto intervenire molto marginalmente sul nostro sistema penale perché le norme erano già contenute nel nostro cui è l'Europa che si è adeguata a ciò che l'Italia aveva fatto - riteniamo che sia necessario completare il lavoro.

per l'istituzione delle squadre investigative comuni sovranazionali - che costituiscono strumenti investigativi comuni ai diversi Paesi per facilitare le indagini e le procedure, specie in questo tipo di reati - possa approdare quanto prima in Aula. Dal gennaio del 2009 il disegno di legge per l'istituzione delle squadre investigative comuni è pronto in Commissione giustizia: che approdi dunque in Aula e dia al nostro Paese lo strumento normativo per contrastare questi fenomeni di criminalità che offendono l'umanità.

la collega Boldi abbia evidenziato a nome della Lega Nord tutti gli aspetti positivi del provvedimento in oggetto. Ricordo inoltre come la Convenzione in esame sia stata firmata dell'Italia ben cinque anni fa, e precisamente in data 8 giugno 2005, e come il presente disegno di legge proponga la sua ratifica in ottemperanza all'obbligo politico di natura internazionale assunto dal nostro Paese all'atto della firma della Convenzione medesima.

ma anche e soprattutto uno strumento efficace ed ineliminabile per tutelare adeguatamente alcuni diritti e alcune libertà fondamentali delle persone. I suoi obiettivi sono la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, sia in ambito nazionale che internazionale, collegate o meno alla criminalità organizzata ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. Il principio fondamentale della Convenzione in oggetto riguarda la protezione e la promozione dei diritti delle vittime, che devono essere assicurati senza alcuna discriminazione di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione,

La Convenzione di Varsavia pone pertanto in risalto il fatto che la tratta costituisce una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all'integrità delle persone e che, in tal senso,

Purtroppo questo fenomeno muove un fatturato miliardario grazie ai profitti derivanti dallo sfruttamento delle persone per fini sessuali, per sfruttamento sui luoghi di lavoro, per accattonaggio, per traffico di organi e per guerre; costituisce quindi un giro di affari che colloca la tratta degli esseri umani al terzo posto nelle attività della criminalità organizzata, dopo la droga e le armi. Il fenomeno della tratta vede coinvolte milioni di persone in tutto il mondo, di cui quasi la metà per sfruttamento sessuale e circa un terzo per sfruttamento economico. Un traffico, quindi, che da un lato porta alla violazione dei diritti umani, da un altro è frutto di un crimine che trae ampi vantaggi dalla violazione stessa. Proprio per il carattere del fenomeno, che implica un'offerta e una domanda, anche l'impegno culturale e la sensibilità per la riaffermazione dei diritti delle persone e della dignità di ogni essere umano dovrebbero essere promossi a tutti i livelli, da quello governativo a quello educativo. In sintesi, quindi, si può ricordare tale atto con la regola delle prevenire la tratta; proteggere i diritti delle vittime; perseguire gli autori del reato, promuovere la cooperazione internazionale. Per ultimo, esprimo l'auspicio ad una corretta applicazione di quanto previsto all'articolo 14 della Convenzione. Infatti, tale articolo giustamente prevede la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno alle vittime della tratta. Questo avviene per due ordini di motivi, per ragioni umanitarie e per consentire la cooperazione con le autorità. Infatti, si prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato se ricorra una o entrambe delle seguenti condizioni: che la permanenza della vittima sul territorio dello Stato parte sia ritenuta necessaria per la collaborazione che può prestare alle investigazioni o ai procedimenti penali, oppure necessaria in considerazione della situazione personale della vittima stessa. la seconda delle anzidette condizioni sia particolarmente rilevante perché, anche in considerazione della genericità con la quale è stata formulata, può consentire il rilascio del permesso di soggiorno anche per ragioni non collegate alla collaborazione con le autorità competenti. La vittima viene in tal caso presa in considerazione in quanto persona che ha subito una lesione nei propri diritti fondamentali e non solo in quanto persona che può fornire informazioni utili per contrastare l'attività dei trafficanti.

sottolineando nel contempo che solo i soggetti vittime della tratta possono essere gli interessati esclusivi di quanto previsto dall'articolo 14 e che non vi siano invenzioni di sorta. Per concludere e per far meglio comprendere il nostro pensiero vorrei rubare una dichiarazione rilasciata dal ministro Maroni circa il rimpatrio dei minori. Il Ministro dice: «Potremmo rimpatriare i minori che vengono da un altro Paese europeo. Questa situazione si verifica talvolta con minori che sui traghetti arrivano direttamente nei porti italiani, ad esempio dalla Grecia o da Patrasso. Ma se sono minori, noi comunque li teniamo in Italia, non li rimandiamo in Grecia, pur potendolo fare». Questo è un altro elemento che caratterizza le buone prassi italiane dal punto di vista dell'accoglienza e dell'integrazione e non solo del contrasto all'immigrazione clandestina. dichiarando pertanto necessario che il nostro Paese ratifichi questa importante convenzione e, conseguentemente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

prendo la parola a nome del Partito Democratico ovviamente per annunciare il voto alla ratifica della convenzione, da noi auspicata fin dalla precedente legislatura e sollecitata nell'attuale con ben tre disegni di legge, che hanno indotto il Governo a presentare finalmente un proprio disegno di legge di ratifica.

presso il cui Dipartimento siede la commissione interministeriale per il sostegno alle vittime della tratta, della violenza e del grave sfruttamento, aveva dichiarato in Senato, rispondendo ad una specifica interpellanza sul tema, che non vi era interesse del Governo alla ratifica. Come già messo in luce in discussione generale, l'Italia è interessata da oltre un decennio dal fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e della prostituzione migrante. seguito del consolidamento dell'esperienza in tale settore, occorre sviluppare azioni tese a contrastare anche le altre forme di sfruttamento, *in primis* quello lavorativo. Tralascio di esporre quali sono le ragioni, che già ho indicato nella discussione generale e che comunque sono nell'intervento scritto, che hanno consentito di far raggiungere all'Italia una particolare maturità

che la Convenzione venga ratificata poiché recepisce la nostra legislazione che deve essere implementata. Negli ultimi anni il fenomeno finora più conosciuto, quello della prostituzione coatta, è profondamente cambiato Potremmo dire oggi che le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico hanno modificato le modalità di reclutamento, di trasporto e di assoggettamento para-schiavistico delle vittime. In sostanza le modalità di reclutamento forzoso sono forme che oggi si presentano come residuali, poiché molto spesso la vittima è consenziente e una volta giunta e una volta giunta nel Paese di destinazione si trova però sottoposta ad una posizione di mercificazione della persona. In altri termini, rimane fermo l'annichilimento, la compressione della dignità, della libertà dell'autonomia e la negazione dei diritti fondamentali Queste trasformazioni non possono essere ignorate anche quando parlamentari e Governo presentano e sostengono disegni di legge in materia di prostituzione. Per questo ci auguriamo che il Governo e la maggioranza desistano dal chiedere al Parlamento l'approvazione dell'Atto Senato n. che, anche se motivato da un diverso intento, dichiarato nella relazione introduttiva, indebolisce il contrasto alla tratta degli esseri umani e criminalizza le vittime. Anche per questo sosteniamo fortemente la ratifica della Convenzione di Varsavia. Aggiungo poi che a queste trasformazioni della modalità di sfruttamento si affianca l'emersione di nuove e preoccupanti forme di schiavitù. II fenomeno dello sfruttamento in campo lavorativo sta diventando sempre più rilevante dal punto di vista sociale ed impone uno sforzo straordinario. I fatti avvenuti in Puglia, in Campania e più recentemente in Calabria, a Rosarno, devono scuotere le nostre coscienze ed imporre a noi legislatori interventi seri, attenti, efficaci. Al riguardo, ricordo che il Partito Democratico ha presentato in Senato disegni di legge che cercano di contrastare in modo emblematico tali gravissimi fenomeni. Richiamo in particolare il disegno di legge Atto Senato n. 753, recante "Norme per il contrasto del grave sfruttamento del lavoro e per la tutela delle vittime", che, presentato a mia prima firma nel lontano giugno 2008, è stato fatto proprio dal Gruppo del PD e che ci auguriamo che venga trattato, discusso e condiviso dalla maggioranza anche nello spirito della Convenzione di Varsavia, che ci accingiamo a ratificare. Devo in ultimo far presente che l'Italia ha una lunga tradizione in materia di contrasto al traffico degli esseri umani e che dovrebbe, quindi, essere in prima fila nel dar seguito al contenuto di tutte le azioni che in Europa e presso le Nazioni Unite vengono portate avanti con determinazione. *(Applausi dal Gruppo del PdL)*. Da ultimo, 1'Italia dovrebbe, solo se il Governo lo volesse, dare piena e completa adesione ed esecuzione alla raccomandazione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta di esseri umani. Con tale raccomandazione, tra l'altro, gli Stati si impegnano a garantire che la lotta contro la tratta di esseri umani rimanga ai primi posti dell'ordine del giorno anche e soprattutto durante i periodi di crisi economica e finanziaria, in fase di elaborazione dei programmi di ripresa. Sempre l'atto del Parlamento europeo prevede che l'assistenza alle vittime sia incondizionata, che l'accesso ad almeno un permesso di soggiorno temporaneo venga rilasciato alle vittime indipendentemente dalla loro volontà di collaborare, che le vittime siano agevolate nel mercato del lavoro, che vi sia accesso a un alloggio adeguato e sicuro, a servizi di supporto specializzato, a servizi di assistenza, traduzione e interpretazione ove necessario per contattare la famiglia e gli amici e che sia garantito l'accesso all'istruzione per i bambini. inoltre, una politica semplificata del ricongiungimento familiare per le vittime, in particolare nei casi in cui ciò sia necessario per la loro protezione e che alle vittime venga fornita assistenza professionale, tra cui una consulenza legale gratuita. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Quanto esposto giustifica ampiamente gli emendamenti presentati al testo dal Partito Democratico e in parte condivisi con colleghi della maggioranza. Si tratta, quindi, di cogliere l'occasione di dar seguito, con la ratifica o con interventi successivi conseguenti, a precise raccomandazioni del Parlamento europeo, perfettamente in linea con la convenzione di Varsavia, che prevede che gli stati membri

Una convergenza della maggioranza su tale misure potrebbe certamente favorire politiche di immigrazione più adeguate, presupposto per un migliore contrasto a tutti i fenomeni illeciti in materia, dal *traffiking* alla tratta. E in ogni caso il Governo e il Parlamento, senza distinzione di appartenenza politica dei propri componenti, dovrebbero esigere che a chi è debole e schiavo venga doverosamente riconosciuto con la legislazione

Presidente, vorrei chiarire che il rispetto non è per me, che pure come parlamentare lo merito, ma per le vittime della tratta di esseri umani. *(Applausi dal Gruppo* *PD).* Ogni volta che parliamo di diritti umani o di diritti ordinari che ai cittadini devono essere riconosciuti con un sistema di giustizia efficiente

In ogni caso Governo e Parlamento, senza distinzione di appartenenza politica dei propri componenti, dovrebbero esigere che a chi è debole e schiavo venga doverosamente riconosciuto, con la legislazione e con i fatti, il diritto di essere rispettato e tutelato nella persona e nella dignità chi è preposto alla lotta al traffico, alla mercificazione, allo sfruttamento degli esseri umani non vengano sottratti strumenti di indagine, ma anzi vengano rafforzati con mezzi di contrasto in campo nazionale, europeo e trasnazionale.

questa complessa strategia è espressa in maniera emblematica dalla Convenzione n. 192 del Consiglio d'Europa, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005 e firmata dall'Italia il ben lontano 8 giugno 2005, che stiamo finalmente per ratificare. *(Applausi

che riguarda una materia particolarmente delicata e che incide su alcune fattispecie di reato che devono trovare un contemperamento di interessi fra le diverse categorie anche produttive interessate a tali fattispecie di reato. Dunque chiedo, se vi è unanimità da parte dei Gruppi, il rinvio alle Commissioni competenti del disegno di legge in esame.

noi abbiamo concordato con l'ipotesi secondo cui, per avere un voto unanime e veloce, perché più volte questa Convenzione doveva essere discussa ed è stata rinviata, sia necessario un ulteriore approfondimento in tempi brevissimi - così si diceva

sono già trattati nell'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento per il codice penale, che contiene già oggi l'esclusione dell'applicabilità della norma penale sul maltrattamento alle attività di allevamento, caccia, macellazione e trasporto disciplinate da norme di settore. Se però - indipendentemente da queste considerazioni, che approfondimenti di queste ore ci hanno consentito di verificare

Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che il testo oggi all'esame dell'Aula fosse già un testo assolutamente coerente con la legislazione oggi vigente. si tratta di una ratifica che il mondo animalista, ma anche il mondo della veterinaria e tutte le persone che hanno interesse verso il mondo degli animali stanno aspettando da tantissimo tempo, perché contiene norme che riguardano non solo il maltrattamento degli animali, ma anche il traffico illecito degli animali, che sappiamo essere un problema molto importante, che si ripete quasi quotidianamente. Detto questo, noi - come dire - non ci opponiamo ad una rimessione in Commissione purché - questa è la nostra condizione qualcuno, non so se il relatore o il Presidente del Senato, ci garantisca che il provvedimento ritorni in Aula entro al massimo due settimane, perché non accettiamo più che questo provvedimento venga rinviato *sine die*. Poiché non si fanno osservazioni, la proposta si intende accolta. È ovvio che sarà compito dei Capigruppo chiedere alla Presidenza di calendarizzare il più presto possibile il provvedimento.

il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, riguarda l'Accordo di sede tra l'Italia e il *Network* internazionale di centri per l'astrofìsica relativistica in Pescara, denominato ICRANET. Ricordo che l'Italia ha aderito dal 2003 all'Accordo istitutivo appunto del *Network* internazionale di centri di ricerca nel campo dell'astrofisica relativistica, sorto sorto nel 1985 per iniziativa dei premi Nobel per la fisica Riccardo Giacconi ed Abdus Salam, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica internazionale. Aderiscono all'intesa anche Armenia, Brasile e Città del Vaticano, sedi di importanti centri di osservazione astrofisica. istitutivo, ratificato con la legge 10 febbraio 2005, n. 31, oltre a qualificare l'ICRANET come «organizzazione internazionale indipendente», dispone che la sede del *Network* sia a Pescara. L'Accordo in esame integra la cornice normativa, assicurando una serie di agevolazioni, già concesse dall'Italia, quale Paese ospitante, ad altri organismi delle Nazioni Unite che hanno sede nel nostro Paese, ad un'istituzione scientifica internazionalmente riconosciuta come una struttura di eccellenza. Nei contenuti, l'articolo 2 stabilisce che il Governo italiano riconosce la personalità giuridica all'ICRANET, e quindi la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni e di stare in giudizio. Ai sensi dell'articolo 3 il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara porrà a disposizione di ICRANET, in via gratuita, il complesso sito in della Repubblica n. 10, già individuato da una Convenzione allegata all'Accordo di sede. In base a tale Convenzione, la città ha concesso in comodato gratuito una sede di circa 1.200 metri quadrati, ristrutturata e munita delle più avanzate tecnologie multimediali. Le spese di manutenzione straordinaria della sede sono a carico del Comune, mentre quelle per la manutenzione ordinaria sono sostenute dal *Network*. L'articolo 4 prevede l'inviolabilità dei locali, degli edifici, dei terreni e degli archivi utilizzati dall'organismo. Il direttore dell'ICRANET si impegna a evitare che i locali possano essere utilizzati come rifugio per persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'estradizione in un altro Paese. L'articolo 5 prevede che i beni e gli averi dell'organismo destinati al perseguimento dei fini istituzionali siano immuni dal procedimento legale e dalle misure esecutive, amministrative o giudiziarie; l'immunità dalla giurisdizione e dalla relativa esecuzione non viene riconosciuta in relazione a danni causati da veicoli, imbarcazioni o aeroplani di proprietà, ovvero utilizzati dall'ICRANET, nonché in relazione a violazioni del codice stradale, nautico o aeronautico, come pure per la stipula dei contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi secondo le disposizioni del regolamento del personale. L'articolo 6 esclude la responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano per le attività svolte dall'ICRANET e dal suo personale sul territorio nazionale; è previsto altresì il diritto di rivalsa nei confronti dell'ICRANET qualora venga fatto ricorso alla responsabilità del Governo italiano. L'articolo 7 reca la responsabilità esclusiva dell'ICRANET per tutti i danni provocati dalle proprie attività in Italia. Si esclude qualsiasi richiesta di risarcimento al Governo italiano per i danni prodotti a terzi, e l'organismo si impegna a stipulare un'assicurazione per la copertura del danno relativo alla responsabilità civile verso i terzi causato nell'esercizio delle proprie attività. È prevista altresì, all'articolo 9, l'esenzione dalle tasse e dalle imposte dovute allo Stato ovvero agli enti locali, relative a beni o redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti e destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'organismo. È stabilita la non imponibilità agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e di servizi di importo «rilevante», cioè superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale (oggi pari a circa 258 euro) per le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia. È altresì prevista l'esenzione dai dazi doganali e dalle imposte sull'importazione e sull'esportazione dei beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ICRANET. Ai sensi dell'articolo 11 sono concessi privilegi e immunità, unicamente per garantire lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET, al personale. L'articolo 12 riconosce il diritto per l'ICRANET di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane, in qualsiasi altra località in Italia. L'articolo 13 disciplina i privilegi e le immunità concesse al personale che partecipa a tali riunioni, ovvero convocato dall'ICRANET, in analogia alle agevolazioni previste per i rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea. Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica il secondo l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 440.000 euro all'anno a decorrere dal 2010. Detti oneri sono essenzialmente correlati alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo sui privilegi e immunità spettanti al personale. La copertura finanziaria del provvedimento risulta a valere sui fondi stanziati in relazione alla Convenzione ONU sulla lotta alla desertificazione. Si tratta della medesima modalità di copertura prevista anche dal disegno di legge n. 1881 recante il Protocollo di modifica della Convenzione tra Italia e Francia sulle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia, già approvato anche dalla Camera dei deputati. Nel corso dei lavori della Commissione sono state fornite assicurazioni da parte del Governo che il combinato disposto dei due provvedimenti non si tradurrà nel sostanziale azzeramento delle citate disponibilità, ma che la Convenzione per la lotta contro la desertificazione verrà rifinanziata, al fine di mantenere inalterato l'importante contributo del nostro Paese alla lotta contro la desertificazione. Auspico pertanto che il Governo voglia tener fede a questo impegno preso con il Parlamento. inoltre che l'adozione dell'Accordo in esame possa produrre positivi effetti sull'intero territorio abruzzese, già provato dal recente drammatico terremoto e si traduca in un sostegno alla ricerca e allo sviluppo dell'industria italiana. Va considerato, infatti, anche il significato simbolico dell'Accordo. L'Abruzzo vantava, con il polo universitario d'eccellenza dell'Aquila, un livello di investimenti nella ricerca assolutamente avanzato rispetto alla media italiana; era cioè capace di attrarre cervelli dall'estero, invertendo il triste fenomeno del nostro Paese che vede i migliori studenti italiani emigrare e nessuno arrivare nelle sedi di ricerca dall'estero. Dopo la tragedia del terremoto, questo Accordo rappresenta il primo passo per ricostruire quella eccellenza, e la scelta di Pescara come sede del centro non è pertanto casuale. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con l'osservazione che in relazione all'attività

È presente in tribuna una rappresentanza di studenti della Scuola media statale «Guglielmo Marconi» di Vittoria, in provincia di Ragusa. A loro va il saluto dell'Aula.

Si tratta di un istituto presente nella mia città, per cui non posso che esprimere un doppio sì a questo provvedimento. Esso conferma una scelta positiva dell'amministrazione comunale che risale a qualche anno fa

***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006***

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. La Commissione osserva tuttavia che il meccanismo di monitoraggio della perdita di gettito IVA derivante dall'Accordo,

a legislazione vigente, né elementi idonei a stabilire l'onere effettivo associato all'originaria disposizione di spesa. Tale tipologia di copertura è sempre più ricorrente e non configura propriamente i requisiti richiesti dalla legge n. 196 del 2009.

DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998

spesa. Tale tipologia di copertura è sempre più ricorrente e non configura propriamente i requisiti richiesti dalla legge n. 196 del 2009. In relazione alla clausola di salvaguardia, concernente la riduzione

professionale che essi stanno svolgendo in quel Paese, sia la presenza di tre italiani all'interno di una struttura che

Io ricordavo, e ho ricordato al ministro Frattini, che dietro questa maglietta c'è l'Italia, c'è il rispetto di un Paese che sta operando per salvare vite umane. Credo sia stato un atto indegno, e mio dovere era quello di portare all'attenzione di tutti i colleghi questo atto veramente vergognoso.

è bene - credo - ad una certa ora del pomeriggio mettere un po' di pepe in una seduta che - ahinoi - non ha portato nessun tipo di approfondimento dei documenti che abbiamo affrontato fino a questo momento. Lo dico perché in passato mi ero riproposto di chiedere sistematicamente il voto elettronico per quanto riguarda i Trattati; questa è la prima seduta dopo il rientro dalle vacanze pasquali e quindi non lo farò.

in virtù dell'articolo 18 dell'Accordo stesso che parla di risoluzione delle vertenze. Sappiamo che l'Accordo - questo non è un Trattato ma è un Accordo - si fa tra Stati sovrani. Nel caso di specie, Hong Kong non è uno Stato sovrano perché, come è stato ricordato all'inizio, fa parte della Repubblica popolare cinese. Se andiamo a vedere qual è il meccanismo insito nell'Accordo relativamente alla risoluzione delle vertenze, si dice che eventuali vertenze sorte dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'esecuzione del presente Accordo vengono risolte per via diplomatica se le autorità centrali non riescono a raggiungere un accordo direttamente. Le autorità centrali sono due enti che verranno creati, uno nel nostro Paese e uno a Hong Kong, per prendere in considerazione tutte le richieste che saranno fatte relativamente alle varie clausole di questo Accordo, che peraltro è molto ben scritto. Allora, se si tratta di una risoluzione di conflitti attraverso le vie diplomatiche, necessariamente i nostri diplomatici dovranno avere a che fare con quelli della Repubblica popolare cinese che,

del diritto e sicuramente, visto e considerato che si parla di questioni penali, anche dei diritti umani. Non so se il Governo ci può tranquillizzare da questo punto di vista, comunque io ritengo di non partecipare al voto, astenendomi

nella *Gazzetta Ufficiale.* DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008

le condizioni dei lavoratori frontalieri e il transito verso l'aeroporto di Malpensa; inoltre, esso non comporta coperture finanziarie perché già pianificato nelle infrastrutture.

generale dei collegamenti per i viaggiatori tra la Svizzera e l'Italia. Da novembre dell'anno scorso sono scomparsi tutti i treni notturni: non si può andare oltre Milano e non ci sono più i collegamenti con città importanti come Roma.

rispetto ad altre forme di trasporto e permette altresì di incrementare l'efficienza dei collegamenti con l'aeroporto di Malpensa, con evidenti ripercussioni positive per lo sviluppo dell'intera area italo-svizzera.

Signor Presidente, una riflessione di tipo generale sul testo di legge che ci accingiamo ad esaminare e a trattare in quest'Aula suggerisce immediatamente l'idea di una tensione fra passato e futuro, fra modernità e vetustà delle strutture degli apparati normativi, competitività di un Paese o ancoraggio dello stesso a retaggi antichi di tipo corporativo, che suggeriscono - volendo evocare una suggestione olfattiva - l'odore di naftalina.

Se ascoltiamo in religioso silenzio il senatore Carofiglio, facciamo cosa utile. Nessuno è obbligato a stare in Aula.

È un testo di legge che si è attirato le critiche di dottrina consapevole, soprattutto dell'Autorità *antitrust* in molti punti, che segna in maniera vistosa dei passi indietro rispetto alla situazione attuale e soprattutto rispetto agli *standard* cui noi dovremmo mirare aspirando al posto che in teoria dovrebbe competerci in Europa e nel mondo, *standard* di modernità. Siamo oggi in una situazione in cui i più importanti studi inglesi si accingono alla quotazione in borsa, al contrario siamo pronti ad approvare norme che, nel migliore dei casi, ci riportano alla prima metà del secolo trascorso. Registro tre punti di particolare criticità in questo testo normativo. Sono quelli che hanno a che fare: con i giovani e con l'accesso alla professione; con il tema del rapporto fra la professione stessa e la modernità, con particolare riferimento al modo di rendere nota l'esistenza degli studi, la qualità dell'offerta, ciò che, con espressione riduttiva, si suole chiamare la pubblicità, ma che in realtà riguarda la comunicazione dell'offerta professionale; con il tema, infine, solo in apparenza settoriale e tecnico, delle tariffe professionali. tratta di tre temi sui quali si registra ‑ a mio modo di vedere ‑ un significativo e non apprezzabile passo indietro rispetto alla situazione attuale, figuriamoci rispetto alla situazione dei Paesi europei più avanzati sul cui piano vorremmo o dovremmo collocarci. È una normativa antieuropea, una normativa che non corrisponde all'esigenza di una modernità evoluta e in evoluzione. Diciamo qualcosa in primo luogo sulla materia dell'accesso alla professione. Mi verrà consentita una notazione che non ha nulla di strategico, ma che enuncia uno dei tratti in qualche modo corporativi, seppure per un dettaglio, di questa disciplina: con questa nuova normativa, un magistrato amministrativo, un consigliere di Stato o di Cassazione, qualcuno che ha amministrato la giurisdizione, che ha deciso e ha provveduto non potrà più essere iscritto negli albi degli avvocati senza

Presidente, sono in controtendenza rispetto ai miei precedenti colleghi - provengo dalla magistratura, come forse qualcuno sa - e sono sempre stato un sostenitore dell'accesso degli avvocati in magistratura, perché sono del parere che lo scambio di esperienze, le commistioni, le ibridazioni migliorino piuttosto che peggiorare la qualità delle offerte istituzionali e professionali. Sarei favorevole a concorsi dedicati per avvocati per entrare in magistratura. Sono favorevole a quello che c'è già nel nostro ordinamento, Sono favorevole a quello che c'è già nel nostro ordinamento, cioè l'accesso di avvocati in Corte di cassazione. Però con questa normativa i magistrati, ove lo volessero, non possono diventare avvocati. È un dettaglio numericamente insignificante, ma in qualche modo enuncia in maniera rumorosa e vistosa uno dei profili - come dire - spirituali di questa riforma. tralasciando questa che è veramente materia di dettaglio e che vale più come metafora che come tema di discussione politica e tornando al tema generale dell'accesso alla professione, siamo di fronte ad un impianto normativo alquanto farraginoso, in cui gli ostacoli vengono moltiplicati senza, a mio modo di vedere, migliorare la qualità della selezione; in cui, in contrario avviso rispetto alle opinioni più evolute e a quelle dell'Autorità

successivo alla laurea, in cui l'effetto finale non sarà che il rinforzo, la maggior rigidità di un sistema che purtroppo già oggi conosciamo, per cui la professione di avvocato è - e sempre più sarà - riservata ai figli d'arte. Ciò non è bello, perché alcune delle energie migliori che potrebbero essere adeguatamente trasferite e utilizzate in un mestiere di libertà quale quello dell'avvocatura saranno, come in passato, più che in passato, costrette a rivolgersi altrove, a fronte di un sistema in cui vi è un lunghissimo periodo, privo completamente di garanzie per i giovani, di tirocinio, anzi di tirocini e di esami e di altri esami e selezioni che, se rende più complicato l'accesso alla professione, non rende migliore la selezione di coloro che alla fine giungono a questo traguardo. Dicevo della comunicazione, della pubblicità, espressione riduttiva che utilizziamo per rendere sinteticamente ciò che pensiamo. Viviamo in una società in cui i profili della comunicazione innervano la sostanza, e non solo la forma, delle cose, definiscono lo statuto di esistenza delle cose; una società nella quale l'uso dello strumento informatico e della rete è elemento strategico per far sapere che le cose esistono. Se non si sa che esistono, semplicemente non esistono. In questa legge, volendo utilizzare un altro elemento simbolico, ciò che ci propone l'esistenza dell'offerta legale è la targa davanti allo studio. Non va bene. Non va bene in un'epoca in cui nei Paesi più evoluti siamo veramente molto, molto oltre. Insisto a dire che, oltre alle forme di tutti i tipi di comunicazione dell'esistenza di variegate offerte professionali, si verificano diverse e più potenti ed efficaci forme di organizzazione, addirittura di distribuzione, del rischio dell'attività professionale. C'è una norma che opportunamente prevede l'obbligo dell'assicurazione, ma la sua operatività viene rinviata *sine die* all'adozione di una non meglio precisata normativa europea, quindi sostanzialmente viene svuotata di significato. Non va bene neanche questo. Così come non va bene il tema,

l'Autorità *antitrust* sottolinea ed evidenzia come l'intervento sulle tariffe professionali, con l'indicazione di minimi inderogabili, sia gravemente nocivo del principio di concorrenza e dunque - in una società in cui il principio della liberalità delle professioni sia realmente inteso - della qualità del servizio offerto, oltre che della possibilità per i giovani accedere in maniera lineare - e non attraverso operazioni di filibusta professionale - ai clienti importanti, vale a dire ai soggetti istituzionali e alle grandi imprese, i più interessati naturalmente a questa materia. Non è un caso, per enunciare ancora una volta uno dei connotati purtroppo neocorporativi di questa legge, che mentre le tariffe professionali minime sono inderogabili,

il principio ispiratore, più o meno esplicito o implicito, di questo dettato normativo sia quello di chi cerca di fermare le lancette dell'orologio, anche se in questo modo l'unico risultato che si ottiene è quello di rompere l'orologio, mentre la società va avanti.

la garanzia dei diritti e della loro tutela giurisdizionale presupponga necessariamente, oltre ad un giudice indipendente, un'adeguata difesa tecnica, addirittura imposta per processi particolarmente delicati come quello penale. Si pensi, nella storia più o meno recente, ai processi contro i capi storici delle Brigate Rosse, in particolare quelli seguiti a Torino dall'avvocato Croce, poi ucciso dalle stesse BR. A dimostrazione del loro rifiuto dell'ordinamento giuridico inteso nel suo complesso e definito borghese, quegli imputati rifiutavano di essere difesi da un avvocato, perché identificavano il sistema giustizia con l'avvocato. Si dovette tentare all'epoca un'interpretazione dei codici tale da poter escludere la necessità della difesa tecnica nel giudizio penale: questa interpretazione - ritengo a ragione - fu rigettata dalla suprema magistratura, perché si riaffermò il principio dell'indispensabilità dell'avvocato in quei processi come in altri. Analogo problema si pone, in maniera devo dire pregnante, per quanto attiene i settori civile ed amministrativo, con le ulteriori e connesse specializzazioni, se si pensa a come siano mutati negli ultimi decenni i rapporti economici e finanziari, a livello commerciale, societario ed economico tra persone, società o gruppi finanziari appartenenti ed operanti all'interno di uno stesso Stato o in Stati differenti: l'internazionalizzazione del sistema giustizia è ormai una realtà. L'avvocato è sì il difensore, prima di ogni altro, del suo assistito, ma nel contempo è in sostanza anche il garante del corretto svolgimento dei procedimenti e concorre quindi con il giudice a fare in modo che ogni procedimento giudiziario si svolga in conformità delle procedure di legge. Dovremmo concordare quindi sulla necessità che l'avvocato, fermo restando il suo principale compito di difensore, svolga in sostanza anche il ruolo di «garante di legalità». Per fare la vecchia figura e la vecchia organizzazione dell'avvocato in Italia non bastano più. Aggiungo che non poche questioni e confronti/scontri che da tempo caratterizzano i lavori del Parlamento, a mio giudizio scaturiscono o sono decisamente influenzati, se non talvolta originati, dalla condizione in cui versa la categoria degli avvocati. Sono presenti nel nostro Paese in numero di gran lunga superiore rispetto agli altri Paesi europei e non appaiono sempre e tutti all'altezza del compito importante loro affidato. È chiaro, quindi, come sia centrale e prioritario dovere dello Stato quello di assicurare al cittadino che gli avvocati iscritti all'albo siano in grado di esercitare al meglio, con rigore e professionalità, la propria delicata funzione, al fine di garantire non solo la migliore tutela giurisdizionale dei diritti degli assistiti, ma anche l'efficace amministrazione della giustizia. La legge forense - lo ha ricordato il Presidente poco fa in apertura dei lavori - è un regio Siamo quindi chiamati a modificare un impianto normativo che nel nostro Paese fu varato nel lontano 1933. C'è la necessità di apportare significativi miglioramenti, una necessità che non può essere ulteriormente procrastinata. È stato in più occasioni ricordato

Pertanto, nella convinzione dell'assoluta importanza della valorizzazione della difesa tecnica ai fini del miglioramento complessivo della qualità della giustizia e della tutela giurisdizionale dei diritti, il Partito Democratico, fin dall'inizio della legislatura,

il diritto alla difesa, valorizzando il ruolo dell'avvocatura all'interno del sistema giudiziario, secondo l'indirizzo sancito dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza di Strasburgo e Lussemburgo. Delle molte proposte innovative avanzate nel nostro disegno di legge, si segnalano in particolare le seguenti: attribuzione al Consiglio nazionale forense della competenza ad approvare il codice deontologico, coordinandone le disposizioni con quelle contenute nei codici di condotta degli avvocati di matrice comunitaria; disciplina delle società professionali tra avvocati come società di persone, con la previsione di norme adeguate a tutela del segreto professionale e dei diritti previdenziali dei soci, sulla riga ormai tracciata a livello europeo, come ricordava poc'anzi il subordinazione della possibilità per l'avvocato di dichiarare il possesso di una specializzazione al previo conseguimento di un titolo di abilitazione specifica, quindi una specializzazione reale, all'esito di un corso apposito; nuova disciplina del tariffario, con previsione di limiti minimi e massimi anche a garanzia dell'assistito; semplificazione delle procedure necessarie al rilascio della procura e alla prova della sua validità, nonché eliminazione dei formalismi eccessivi previsti per la sostituzione processuale, che non siano effettivamente funzionali alla tutela dei diritti dell'assistito e del regolare svolgimento del processo; nuova disciplina dell'accesso all'Albo degli avvocati, con la previsione di un elenco speciale per coloro che svolgano attività incompatibili con la professione e debbano quindi sospenderne temporaneamente l'esercizio (principio delicato sul quale tornerò alla fine di questo intervento); subordinazione del rilascio dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al previo superamento di un esame teorico e pratico, con la previsione del necessario ed effettivo svolgimento del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori quale requisito indispensabile per la conservazione dell'iscrizione all'albo speciale; previsione dell'aumento del numero dei componenti degli organi consiliari, al fine di consentire loro di svolgere al meglio le nuove funzioni attribuite (ad esempio, il controllo della formazione permanente degli iscritti, che si aggiunge al controllo sul tirocinio e sulle modalità con cui esso viene svolto); valorizzazione del merito e della effettiva preparazione teorico-pratica del tirocinante ai fini dell'accesso alla professione; nuova disciplina dell'esame di abilitazione con una preselezione per test e una maggiore selettività delle prove; nuove norme in materia di procedimento disciplinare (altro aspetto quanto mai delicato), con l'attribuzione della competenza, relativamente al giudizio disciplinare, a commissioni distrettuali (che in tal senso sostituirebbero i consigli dell'ordine nel controllo disciplinare), le cui decisioni possono essere impugnate dinanzi al Consiglio nazionale forense. La pronuncia di tale organo sarà infine appellabile (come avviene oggi) dinanzi alle sezioni unite della Cassazione. Come già accennato, talune parti di questo nostro disegno di legge sono state sostanzialmente recepite dal testo approvato dalla Commissione, con particolare riferimento ai profili relativi all'adempimento degli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti; all'iscrizione all'albo degli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza; a talune specifiche prerogative del Consiglio nazionale forense; alla nullità degli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia; alla sostituzione in udienza; alla sospensione dall'esercizio professionale; alla cancellazione dall'albo; all'applicabilità ai praticanti delle norme disciplinari previste per gli avvocati; alla frequenza dei tirocinanti alle udienze. Se sotto questi profili dunque può certamente condividersi - e lo condividiamo - il lavoro del Comitato ristretto e della Commissione, sotto altri aspetti esso è decisamente carente e non coglie alcuni dei propositi di riforma suggeriti dal PD, che sono tuttavia necessari per migliorare davvero la qualità del sistema-giustizia, con particolare riferimento ai temi della retribuzione per i tirocinanti, dei minimi tariffari, del sistema delle incompatibilità, della valorizzazione del merito e della ridefinizione dell'esame di abilitazione. Sono tutti punti cruciali e caratterizzanti, sui quali torneremo ad offrire il nostro contributo attraverso gli emendamenti. Pensiamo a quanto sia delicato il tema della corretta definizione delle incompatibilità. È un *punctum dolens*, ma i colleghi della maggioranza, soprattutto coloro i quali hanno maggiore sensibilità ed esperienza anche per aver praticato e continuare a praticare l'attività forense, dovrebbero riflettere con molta serenità. un avvocato che acceda al ruolo ed alle funzioni di parlamentare, se non addirittura di componente del Governo, che vada nelle Commissioni parlamentari o interparlamentari, ovvero che assuma il compito di presiedere organismi economici, finanziari o di alta dirigenza di strutture pubbliche regionali o nazionali. Compiti questi che comportano un potere ed una capacità da porre l'avvocato in una condizione di obiettiva, potenziale possibilità di influenzare il corso regolare dei procedimenti, quando nello stesso tempo egli svolga la duplice funzione. Mi rendo conto che tocchiamo punti delicati e interessi di particolare rilievo ma dobbiamo farlo, amici della maggioranza. Così come si sarebbe dovuto riflettere con maggiore attenzione in ordine ai rischi che comporta, sul piano generale, la mancata previsione di un adeguato sistema di incompatibilità: le troppe leggi *ad personam* non sono forse il frutto della ormai consolidata commistione tra il ruolo di avvocato e quello di parlamentare? Consentitemi la franchezza. Lungi da me la benché minima intenzione di sfiorare solamente la rispettabilità dei colleghi interessati, ma vi chiedo: non percepite alcun disagio nel momento in cui avvocati difensori in piena attività, come difensori per esempio del Presidente del Consiglio dei ministri o di altri eminenti e potenti personaggi del sistema politico-istituzionale del Paese, svolgendo le funzioni parlamentari, presentino e sostengano in Aula o nelle Commissioni disegni di legge che servono innanzi tutto ed immediatamente - anche se non in maniera esclusiva - a risolvere problemi inerenti a processi in pendenza o a carico proprio dello stesso *Premier* o di altri potenti suoi collaboratori? Sono questi i profili che il disegno di legge non ha il coraggio di affrontare e che pertanto non ci consentono di condividerne appieno l'impianto, nella convinzione che il tema della riforma dell'avvocatura sia un tema centrale per la giustizia su cui si gioca una sfida per il Paese, che trascende le sole categorie professionali direttamente interessate, per coinvolgere invece la generalità dei cittadini e l'effettività della tutela dei diritti. Per queste ragioni, noi ci rivolgiamo alla maggioranza di Governo affinché rifletta e perché non si perda questa grande occasione storica di una riforma che sia veramente tale ed adatta a soddisfare gli interessi superiori della giustizia nel nostro Paese. a disposizione venti minuti, ma non è che sono un caso singolare: è una delle poche occasioni in cui quest'Aula si trova a discutere senza avere i tempi contingentati, quindi ciascun senatore può liberamente intervenire fino ad un tempo massimo di venti minuti. Non bisogna essere obbligatoriamente prolissi, anzi, la sintesi spesso è un buon dono; ciò non vuol dire che se occorre se occorre argomentare maggiormente le proprie tesi e vi sono motivazioni che spingono ad intervenire, credo che questa sia una delle poche occasioni dove il non contingentamento dei tempi dà a quest'Aula l'occasione di essere davvero Parlamento, nel senso di poter parlare ed intervenire sull'argomento. riforma dell'ordine forense. Riforma forse è una parola che mal si addice al testo che andiamo ad esaminare; controriforma forse già potrebbe essere più idoneo come termine. Perché dico controriforma? L'accenno alla data del testo che andiamo a rivedere ormai lo abbiamo già fatto.

si tutelano ulteriormente i consumatori, quelli che poi si rivolgono agli avvocati. La Spagna ha delle leggi del 1995, ma interviene anche nel 2001 con lo statuto generale dell'avvocatura spagnola;

e gestire la società dei fasci e delle corporazioni e, in qualche modo, di indirizzarla. Nel 2010 abbiamo una situazione praticamente inversa, dove i fasci e le corporazioni - in questo caso gli ordini

non ricordo sia mai avvenuto prima. Addirittura il Consiglio nazionale forense, l'organo istituzionale più alto dell'avvocatura, ha ritenuto doveroso e opportuno - questo ci lusinga molto prendere una intera pagina di grandi quotidiani a tiratura nazionale per dire che il documento licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, riguardante il nuovo ordinamento forense, è apprezzabile e condiviso, un documento del quale si auspica la celere definizione. Reputo questo un motivo di grande soddisfazione». Io, invece, non reputo motivo di soddisfazione il fatto che un ordine ci consegni un testo e noi, come Parlamento, lo prendiamo, lo recepiamo e ne facciamo una legge.

trova anche un buon riassunto su come Inghilterra, Galles, Spagna, Francia e Germania affrontino i punti nodali che sono già emersi fino ad oggi.

È così che si tutela un cittadino che ri rivolge ad un avvocato e che vorrebbe avvalersi di un buon professionista? Come fa il cittadino a scegliere, in un mercato così organizzato, il buon professionista?

La Commissione lavoro su questo tema davvero non esiste? La professione dell'avvocato non può essere affrontata anche come professione, come lavoro? È È un'entità astratta che deve essere esaminata nella sola Commissione giustizia? L'Autorità *antitrust* vi ha mandato una serie di osservazioni lunghissime e approfondite,

che viene presa in considerazione solo se esprime un parere conforme a quello della maggioranza e del Governo? Credo che la sua inutilità sarebbe davvero scritta. Abbiamo trasformato

gli appunti che fa l'*Antitrust* sull'accesso alla professione, sul Consiglio nazionale forense e su quanta potestà di regolamentazione è rimasta in capo ad esso, sulle associazioni sulle associazioni multidisciplinari, sulle incompatibilità, sulle tariffe, sulla pubblicità, sulle specializzazioni e sulle rigidità ancora una volta del Consiglio nazionale forense.

Non sono particolarmente ottimista, anche perché sappiamo bene che domani, proprio al Ministero della giustizia, sono stati organizzati gli stati generali delle corporazioni. È una definizione forse un po' si tratta, degli stati generali degli ordini professionali e quindi delle corporazioni. Tra l'altro, colgo l'occasione per ricordare che domattina alle ore «Radicali italiani» organizzerà un presidio proprio davanti al Ministero della giustizia contro gli stati generali delle corporazioni, perché le professioni siano davvero libere.

come segnalava il relatore Valentino, è d'accordo sul disegno di legge in esame. Anche se il Consiglio nazionale forense ha avuto il buon gusto di spendere dei soldi per fare pubblicità

do questa informazione, che non vuol significare che bisogna fare una legge scritta su Facebook: credo tuttavia che anche questi siano appunti utili al dibattito e alla discussione, e che le pagine del Consiglio nazionale forense non rappresentino tutta l'avvocatura e tutti i professionisti.

sta nell'articolo 2, quando si prevede: "L'iscrizione a un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato". È quindi l'iscrizione all'albo che dà titolo per esercitare, non l'avere studiato all'università studiato all'università ed avere superato l'esame di Stato. È l'ordine che dà la patente per potersi dire avvocato. Si va avanti nell'assurdo quando, all'articolo 22, si legge: «Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza...». Come si fa a pensare che un'associazione di avvocati abbia come finalità prevalente quella di tutelare tutelare tutti gli altri, tutti quelli che non sono iscritti a quell'ordine? È normale che un ordine, un'associazione, una corporazione tuteli i propri iscritti;

finestra"). Onorevoli colleghi, come già comunicato ai Gruppi per le vie brevi, la seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 10,30, anziché alle ore 9,30, come precedentemente stabilito.